come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, do ora la parola, per cinque minuti ciascuno, ai senatori che desiderano intervenire sul grave episodio di violenza che ha interessato una famiglia di origine pakistana a Novi di Modena.

Tutti noi abbiamo saputo che un cittadino pakistano ha ucciso la moglie a sassate perché ha osato difendere la volontà della figlia di rifiutare un matrimonio combinato dal padre con un uomo a lei non gradito. Tutti noi abbiamo saputo che contestualmente il fratello di Nosheen ha tentato l'uccisione della sorella a sprangate per dimostrare la determinazione del fondamentalismo a sostenere che il libero arbitrio, che la volontà di decidere della propria vita, non è un diritto riconosciuto, per le donne. Ho detto bene: per le donne non è un diritto riconosciuto. Tutti abbiamo preso atto che il Ministero per le pari opportunità si è costituito parte civile nel processo che seguirà a questo terribile doppio reato, iniziativa assunta anche per Hina e per Sanah, ragazze perfettamente integrate nella società civile del nostro Paese, ragazze che avevano maturato la consapevolezza delle grandi opportunità che il nostro Paese offre in termini di integrazione e di successo personale nel mondo lavorativo e sociale. Per questo hanno subito, nel nostro Paese, una condanna a morte per nome e per conto di una religione integralista che si permette, attraverso un ramificato e silenzioso quanto terribile senso di appartenenza ed obbedienza, di mettere in atto ciò che è contro la nostra legge. La nostra Costituzione sancisce l'uguaglianza tra uomo e donna, sancisce le pari opportunità tra uomo e donna, sancisce che ogni persona può e deve contribuire al benessere della Nazione, sancisce che ciascuno può disporre della libertà di scelta in campo personale e professionale nel rispetto delle leggi. La nostra Costituzione condanna la pena di morte. la nostra Costituzione condanna la pena di morte. Per quanto mi riguarda, affermo con forza che le vittime dell'integralismo non sono figlie di nessuno. Hina, Sanah e Nosheen appartengono a tutti noi e noi abbiamo il dovere di difendere il positivo messaggio di libertà che ci hanno inviato e per il quale hanno pagato pesantemente. Mi auguro che Nosheen superi il dolore fisico e psicologico subito, con la stessa forza con la quale ha difeso la propria libertà. La Lega Nord da sempre dice che integrazione non è solo lavorare onestamente nel nostro Paese; la Lega Nord ha sempre sostenuto che integrazione significa anche lavorare per implementare, nei cittadini stranieri, il senso delle istituzioni, il senso di appartenenza nella condivisione dei valori che sono alla base del nostro ordinamento giuridico, del nostro «respirare» quotidiano la libertà sancita per ogni persona. Ecco perché abbiamo sempre sostenuto che chi non accetta tutto ciò è bene che torni a casa sua. Non accettiamo, qui, coloro che minano la sicurezza personale, che offendono la sensibilità dei cittadini, che non accettano le nostre leggi, che applicano la pena di morte sfidando tutti. La Lega Nord vuole anche porre l'accento sull'atto di eroismo della mamma di Nosheen che ha dato la vita per difendere le istanze della figlia, le nostre istanze. Dobbiamo riconoscerle che è stata capace di dimostrare a tutti che ci sono donne che, nonostante tutto, alla fine sanno ribellarsi, anche a costo della vita, a ciò che è fuori dalla ragione, alla cruda e gratuita violenza. Ha indicato a tutti noi, questa donna, questa mamma, col sacrificio della sua vita, senza alcuna ipocrisia, senza se e senza ma, qual è la vera strada dell'integrazione dei cittadini stranieri nel nostro Paese.

perché difendeva la figlia che rifiutava un matrimonio imposto dal padre-padrone. Ora Begm Shnez è morta e la figlia Nosheen è in coma. L'Italia non è il Pakistan. Il delitto d'onore non è tollerato. Purtroppo, invece, siamo ancora una volta di fronte al dramma di una integrazione totalmente fallita, se pensiamo che questa famiglia risiedeva qui da almeno dieci anni e non aveva problemi economici. È solo l'ultimo di tanti, troppi casi di tragedia culturale: il fenomeno sta emergendo in tutta la sua drammaticità, proprio a causa della diffusione di episodi che non risparmiano nemmeno che non risparmiano nemmeno altri Paesi europei. Questi delitti d'onore altro non sono che la punta di un iceberg che non riusciamo a vedere perché, della totalità delle donne islamiche che vivono nel nostro Paese, solo pochissime hanno la forza o la possibilità di opporsi ai soprusi. Non devo sicuramente ricordare gli altri due casi, quello di Hina e quello di Sanah, lo stesso uccise perché rifiutavano un matrimonio imposto e tentavano di integrarsi nel Paese che le ospitava: sappiamo benissimo che all'interno di alcune culture orientali il matrimonio combinato è quasi la norma, così come lo era nel nostro Paese, e soprattutto nel Sud, cento anni fa, quando le usanze costringevano le donne ad un ruolo assolutamente marginale. In questa particolare e intollerabile tragedia femminile vi è, tuttavia, un passaggio da non sottovalutare - ripreso anche dalla senatrice Aderenti - in quanto segnale importante di un cambiamento in atto: vi è una donna che si è ribellata al marito per difendere le ragioni della figlia. La vittima non voleva che la figlia avesse una relazione infelice come quella che lei stessa era stata costretta a vivere. E allora, affinché la sua morte non sia stata vana, è ora di passare all'azione con politiche rigorose. Che fare? L'antidoto è l'interazione tra culture che, al di là della via normativa, è sicuramente capace di produrre il mutamento culturale. Delitti come questi saranno tanto meno frequenti quanto più la società italiana riuscirà a definire una convivenza in cui i diversi gruppi etnici e religiosi presenti nel nostro territorio entreranno in contatto tra loro. L'alternativa è la chiusura etnica, il riprodursi di culture ostili l'una all'altra; insomma, il peggio, del quale le prime vittime saranno sempre le donne. Ed ancora, associandoci all'appello dell'onorevole Sbai, vorrei chiedere al ministro dell'interno Maroni di intervenire sul Comitato per l'Islam italiano del Viminale affinché velocizzi l'*iter* per aprire l'albo degli imam e avviare un censimento delle moschee in Italia perché, se davvero il pakistano che ha ucciso la moglie è il proprietario della moschea locale, ciò dimostra la pericolosità delle moschee fai da te. Bene ha fatto il ministro Carfagna a chiedere di potersi costituire parte civile nel processo contro Ahmad Khan Butt perché ciò rappresenta lo sdegno di tutto il nostro Paese e la nostra fermissima condanna ad ogni atto di violenza. Chi compie violenza contro le donne ed addirittura pensa di disporre della loro vita non deve trovare accoglienza nel nostro Paese. Non ci sono alibi né scusanti. *(Applausi del senatore italiano o no, si macchi di questo genere di reati. Dobbiamo in tutti i modi convincere le giovani straniere che stanno costruendo in Italia il loro futuro a denunciare ogni sopruso, liberarsi appena possono e farlo prima che si verifichino tragedie come queste. Io stessa ho recentemente presentato un disegno di legge che vieta in maniera totale l'uso di indumenti a copertura del volto, indossati in luoghi che non siano abitazioni private. Certamente l'approvazione veloce di una legge che vieta il *burqa* ed il *niqab* sarebbe già un gesto concreto nei riguardi di quanto gli italiani ci chiedono. Sarebbe un primo passo, ma la speranza è anche che sia uno stimolo per le donne ad avere coraggio e determinazione, ricordando loro che anche nel nostro Paese, fino a pochi decenni fa, c'erano dalle mie parti donne che andavano col capo coperto da un velo nero.

ha ucciso il proprio figlio appena nato. Credo che tanti altri fatti criminali e tragici, come quello di Modena e di Trento, e le le statistiche purtroppo incomplete in base alle quali solo nel 2008 sono state assassinate 147 donne, 181 nel 2006 più di 600 tra il 2006 ed oggi, così come tutti i fatti che riguardano che riguardano extracomunitari che delinquono nel nostro Paese ci debba fare riflettere, ma debba al contempo evitarci la confusione. La confusione,

È vero. Nel nostro Paese esiste un problema di integrazione, come esiste un problema di immigrazione, regolare ed irregolare. Questo tema, però, non lo si affronta individuando come modello in negativo di un'integrazione i fatti criminali che si possono verificare. L'analisi che dovremmo fare è più complessa. Se la risposta che diamo a un tema come questo prende che ha in tutti noi determinato profondo sgomento e orrore, di due uomini che uccidono e tentano di uccidere due donne, allora è evidente che tutto questo ci porta fuori strada. Infatti, se di mancata integrazione si deve parlare è perché in questo Paese politiche di integrazione, da parecchi anni, forse da sempre, non se ne sono fatte

al tema dell'integrazione: quella di rispondere con la paura, con l'alzata dei muri, con la repressione a ogni costo, anche quando questa non è necessaria,

che vengono nel nostro Paese, e vengono certamente il più delle volte per esigenze di lavoro e di integrazione temporanea. Anche qui dovremmo distinguere tra l'integrazione *tout court* e quella di chi viene solo per lavorare. allora di evitare discorsi che, alla fine, servono magari ad alimentare la pancia di coloro che immaginano che il problema con lo straniero sia quello di chiudere ogni tipo di rapporto, quasi che questo fosse oggettivamente possibile,

di soluzione per queste situazioni e questi episodi, e trovo anche un po' di superficialità nell'affrontare l'argomento passando, come diceva appunto il collega D'Alia, direttamente a parlare alla pancia di fronte alla commozione e all'orrore. Facili peraltro sono state anche le analogie con il caso di Hina, uccisa quattro anni fa dal padre, sempre pakistano e sempre per motivi familiari legati ai tribalismi etnici dei matrimoni combinati. Non possiamo però confondere questi fenomeni con l'Islam,

Lì è un problema di ordine pubblico, di controllo del territorio, di un centro di permanenza, identificazione e espulsione che non viene realizzato in Veneto, per cui non si riesce a prendere gli irregolari e a trattenerli perché non abbiamo ancora un luogo, dopo che già dal programma del 2001 si parlava di progettarne uno (parlo del Governo Berlusconi del 2001). Lì la soluzione è di ordine pubblico;

per i gravissimi fatti di Novi: il cordoglio per la morte della mamma Begum Shanhaz, la solidarietà alla giovane figlia Nosheen, selvaggiamente picchiata dal fratello perché rifiutava un matrimonio combinato. A lei porgiamo gli auguri di una guarigione il più possibile veloce e vogliamo affermare, così come hanno fatto il Presidente della Regione Emilia-Romagna e le istituzioni locali, che non la lasceremo sola nel suo difficile percorso di ritorno alla vita. I fatti tragici di Novi non vanno strumentalizzati e non vanno affrontati con nessuno spirito di tolleranza, ma con nessuna demagogia. Ci insegnano molte cose. Innanzitutto, ci confermano che dalle donne, dalle ragazze, italiane e immigrate, viene, nel nostro Paese e nel mondo, la forza per imprimere cambiamenti culturali nella società. Ma questa determinazione, quella che Nosheen (la ragazza picchiata selvaggiamente) ha dimostrato per far valere il proprio punto di vista, le proprie scelte, i propri diritti è stata pagata ad un prezzo troppo caro da lei e da tante donne.

così come in tanti altri Paesi del mondo, la prima causa di morte per le donne dai 16 ai 44 anni sono gli omicidi in ambito domestico e che in Italia ogni due giorni viene consumato un delitto in famiglia: 181 donne sono state uccise lo scorso anno ed il 70 per cento di questi delitti (che avvengono uno ogni due giorni) sono rivolti contro le donne; gli altri, troppo frequentemente, nei confronti dei bambini. Queste drammatiche vicende ci dimostrano che la violenza contro le donne è un dato assolutamente troppo forte nel nostro Paese e che troppo poco si fa per prevenirla e per ostacolarla; ci dimostrano anche la problematicità dei temi dell'immigrazione, la particolare sofferenza che accompagna le donne nell'immigrazione, molto delle quali non la scelgono, ma sono costrette a seguire la famiglia spostandosi dai Paesi di origine nel nostro Paese. Ci dimostrano, inoltre, come le nuove generazioni si sentano sempre più italiane e come questo determini delle forti conflittualità

essere la strada giusta per farlo. L'isolamento può solo favorire l'accentuarsi della sopraffazione e delle violenze, in cui le donne sono vittime proprio perché sono portatrici del cambiamento. Faccio un'ultima proposta concreta perché non dobbiamo parlare solo che i fatti siano accaduti: abbiamo bisogno di maggiori servizi che accompagnino e ascoltino le voci di aiuto che vengono dalle donne e dalle famiglie. Mi riferisco, ad esempio, alle reti di solidarietà e alle associazioni tra le donne, ai centri antiviolenza, che ci sono e sono nati

troppo spesso e troppo drammaticamente riguarda tutte le donne nel nostro Paese. Ci riguarda anche quella degli altri Paesi: non a caso, siamo tutti mobilitati per salvare la vita di Sakineh.

Signor Presidente, anch'io desidero innanzitutto esprimere il mio cordoglio per la morte di questa donna pakistana che ha avuto il coraggio, insieme alla figlia, di ribellarsi ad imposizioni lesive della libertà e della dignità della persona. Desidero esprimere poi la mia solidarietà, e quella di tutto il Gruppo dell'Italia dei Valori, a quella ragazza oggi in coma, ferita a sprangate dal fratello, quale auguro di guarire presto e di poter ricominciare a vivere liberamente secondo il proprio volere, anche se sappiamo che non sarà facile superare il trauma vissuto, che sicuramente lascerà un segno indelebile. Non è il primo caso cui assistiamo in Italia, e certamente dobbiamo essere fermi nel condannare e reprimere pratiche che implicano sopraffazione e violenza nei confronti di donne e bambini, la parte più debole delle comunità di stranieri ma anche, spesso la parte più aperta e disponibile all'integrazione. La presenza di un numero sempre maggiore di immigrati ha reso le nostre società multietniche e multiculturali. La prevenzione, di pari passo con l'integrazione, è essenziale; richiede istruzione, conoscenze e confronto; richiede la costituzione di reti e di partenariati, nonché lo scambio di buone pratiche, al fine di eliminare attitudini e quei comportamenti rituali o tradizionali. L'ignoranza - nel senso di ignorare, non conoscere - rappresenta il peggior nemico del progresso culturale e dell'abbattimento di talune barriere la cui origine risiede più nell'indottrinamento che in una reale volontà di seguire determinate raccapriccianti tradizioni. Per quanto condivisibile l'iniziativa del ministro Carfagna di costituirsi parte civile nel processo contro l'uxoricida, è evidente che ciò non basta. Finché nella cultura della maggioranza sarà prevalente la visione repressiva nei confronti di tutti gli immigrati, di chiara matrice leghista, anche chi proverà ad integrarsi resterà comunque solo. Serve invece, come in altri Paesi europei, uno specifico dipartimento per l'integrazione, altrimenti gli immigrati resteranno sempre di più rinchiusi nei loro ghetti e ai margini della nostra società. Il Governo, e il ministro Carfagna in particolare, non possono ricordarsi degli immigrati solo quando accadono tragedie ma devono dare vita a politiche di vera integrazione, affinché chi si trova a vivere situazioni come quella della moglie e della figlia di Ahmad Khan Butt possa non sentirsi solo e sapere di far parte di una società pronta a difenderla efficacemente da pratiche illegali e violente, che devono rispondere solo al codice penale e niente hanno a che vedere con il rispetto delle tradizioni culturali. Per inciso, voglio ricordare alla senatrice Vicari e all'onorevole Santanchè che in Italia non servono leggi demagogiche lettera. È necessario piuttosto che quanto accade ad ogni singola donna, che sia italiana o straniera, ci riguardi. Certamente la nostra voce oggi sarebbe più limpida se si fosse alzata con la forza necessaria in quest'Aula tutte le volte che una donna sia stata vittima della violenza di un uomo. infatti, peggior insidia per la difesa dei diritti umani della pratica dei due pesi e delle due misure. Ci piacerebbe che il Ministro per le pari opportunità si costituisse parte civile ogni qualvolta si verifichi una qualsiasi violenza contro le donne.

una condanna unanime dei gravi episodi di violenza; ci deve essere un impegno perché si rimuovano determinate condizioni dalla vita della nostra società. Sono anche d'accordo - penso lo siamo tutti - sul fatto che la Costituzione è il punto di riferimento irrinunciabile. È nella Costituzione che sono affermati i diritti fondamentali dei cittadini, l'uguaglianza tra uomo e donna, e i processi di integrazione devono svolgersi all'interno dei principi stabiliti dalla Costituzione, non a prescindere dalla stessa. i nostri diritti e i nostri doveri. Sono tuttavia d'accordo (voglio sottolineare anche questo aspetto, come ha fatto nel suo intervento tra gli altri anche il senatore Saia) che è sbagliato invece, e non vero, vero, attribuire episodi di violenza gravissimi, che vanno condannati e sanzionati penalmente e culturalmente, ad impostazioni religiose, alla religione; non è così. Del resto, proprio la senatrice Vicari ricordava che, non secoli fa, ma qualche decennio fa, in Italia esistevano leggi che prevedevano attenuanti quando si compivano delitti d'onore. Quindi, quello che abbiamo di fronte è un impegno per far progredire il cammino della

Viene da una ferita gravissima. Uscirà da un trauma gravissimo. Ha una famiglia sconquassata. Bisogna che le istituzioni le siano vicine perché la sua vita non sia compromessa».

in Francia gli imam parlano francese. È giusto che ci sia un Islam europeo, un Islam italiano e che gli imam siano formati in Italia, senza rappresentare altri Paesi. che nelle moschee si parli italiano; ma per fare questo abbiamo gli strumenti. Lo strumento non è il disinteresse, gli strumenti non sono le pregiudiziali: lo strumento è dato dalle politiche attive. La Costituzione consente

in Parlamento, proprio al Senato e ancora non procedono - sono previsti gli strumenti per affermare le fondamentali scelte che possono aiutare a far vivere le varie culture e le varie religioni all'interno dei principi sanciti

e della Presidenza del Senato sulle inaccettabili parole pronunciate dal senatore Ciarrapico in occasione del dibattito della scorsa settimana Lo faccio a nome del Partito Democratico perché, fino ad oggi, non sono ancora giunte dal presidente Berlusconi e dal presidente Gasparri parole di chiara e netta condanna delle frasi ingiuriose e antisemite udite in quest'Aula. Solo ieri il presidente Schifani ha sentito il dovere di pronunciare parole forti e chiare in proposito. Era tempo e, comunque, lo ringraziamo. Ma non sono ancora giunti i necessari provvedimenti disciplinari previsti, in questi casi, dal nostro Regolamento agli articoli 66 e 67. Riepiloghiamo brevemente i fatti. Dopo la frase del senatore Ciarrapico: «I finiani hanno già ordinato le *kippah*», il presidente di turno, senatore Nania, ha taciuto, incomprensibilmente. Il presidente Berlusconi nella sua replica ha usato la figura retorica dell'amico che sbaglia, ribadendo la storica amicizia verso lo Stato di Israele, che nulla c'entrava con la discussione. Capisco: una maggioranza barcollante ha bisogno di voti, adesso e alle prossime elezioni, e così non si va per il sottile e pazienza se il senatore Ciarrapico usa espressioni xenofobe, o se l'alleato Storace non ha chiaramente superato il passato neofascista. Ma così non va, non può andare. Altrove - si guardi all'esempio di Chirac, a suo tempo in Francia nei confronti del Fronte Nazionale di Le Pen - la destra costituzionale pone sempre paletti chiari nei confronti del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo. Noi invece abbiamo solo le mezze scuse dell'altro ieri del senatore Ciarrapico, che «non valgono nulla», come ha scritto, in una lettera al «Corriere della Sera», Riccardo Pacifici, presidente della Comunità ebraica di Roma. Il senatore Ciarrapico dice di aver voluto solo attaccare Fini e di aver utilizzato a questo scopo un'immagine sbagliata, una semplificazione. Forse, temo, la verità è un'altra: il suo super io non ha sorvegliato le sue parole e così è emerso dal profondo il suo vero profilo, diciamo così culturale, intriso di volgarità veterofasciste e di pregiudizi razziali. Non bastano le mezze scuse di ieri. Chiediamo al collega Ciarrapico - mi spiace che non sia presente in Aula - di fare un passo indietro, di chiedere scusa, non tanto a Israele, quanto agli ebrei italiani e a tutti gli italiani. Non c'entra nulla, infatti, l'amicizia o meno con Israele. Qui sono in gioco i valori costituzionali di tutti gli italiani, a qualunque fede appartengano.

disattenzione nei confronti di una questione importante per il Senato e non solo per i lavori di questa Assemblea. Non vogliamo, infatti, un processo. Non era questa l'intenzione quando ho chiesto la parola. Intendiamo riaffermare i valori costituzionali e l'impegno comune nella lotta contro tutte le intolleranze. Le battute contro gli ebrei fanno infatti parte di quei pregiudizi (come quelli contro i rom, gli omosessuali e tutte le minoranze) oggetto allora, 70 anni fa, di feroce persecuzione, e oggi di tentativi ripetuti di discriminazione. Sono i moderni *idola tribus* della nostra società contemporanea, di cui dobbiamo liberarci al più presto se vogliamo difendere e rafforzare la democrazia nel nostro Paese. Per queste ragioni - mi rivolgo al presidente Gasparri - condividiamo la proposta che i giovani ebrei italiani le hanno avanzato, di sanzionare come Gruppo PdL il senatore Ciarrapico. Lei non può rispondere, balbettando, un "vedremo", "discuteremo". Colga l'occasione anche oggi per ribadire che il PdL è un fermo difensore dei diritti umani e dei diritti di libertà e che non può accettare che un suo membro pronunci frasi antisemite. Per questo chiedo al presidente Schifani non solo di riaffermare le parole che ha già pronunciato qui in Aula, ma anche un provvedimento di censura che chiarisca al Paese che nel Parlamento italiano, sui grandi valori costituzionali, non si transige e men che meno si può scherzare. Mai! qualche giorno fa il senatore Ciarrapico ha affermato, nel corso del dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Berlusconi qui in Senato,

testualmente: «Signor Presidente, 35 parlamentari che non sarebbero mai stati eletti se non li avesse fatti eleggere lei. Torneranno nell'ombra, come nell'ombra tornerà il titolare di quella terza carica dello Stato che ella molto generosamente gli aveva affidato. Fonderà un partito, speriamo che abbia già ordinato le *kippah* con le quali si presenteranno. Perché di questo si tratta: chi ha tradito una volta tradisce sempre.

Ora, non intendo commentare frasi e dichiarazioni - si commentano da sé - che non hanno giustificazioni e per le quali non sono ammesse giustificazioni, ma delle quali bisogna solo scusarsi. E bisogna farlo nelle sedi proprie, cioè dove è avvenuto il fatto: in Parlamento. È come per le barzellette: quelle di pessimo gusto

in questa circostanza il primo a doversi scusare in quest'Aula sia il senatore Ciarrapico, e poi il Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà, che con il suo applauso ha condiviso le parole infami - queste sì, infami Queste sono le ragioni per le quali, signor Presidente, ritengo che sia opportuno chiudere questa vicenda, per sanare una ferita che obiettivamente si apre nelle istituzioni ogniqualvolta si pronunciano parole improprie che, per carità, possono scappare a tutti - siamo tutti esseri umani

attraverso scuse pubbliche istituzionali che rendano ancora più forte e prestigioso il Parlamento e chi in questo Parlamento ci sta per conto degli italiani. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi curerò degli insulti, né di chi li ha lanciati: non meritano una polemica personale. Sono i concetti che mi preoccupano. Mi preoccupa che nel 2010 si usino ancora termini, espressioni e un modo di pensare che ci riportano indietro di 66 anni. È stata usata più volte l'espressione "rinnegati", un termine entrato nel lessico della politica con i seguaci dei totalitarismi fascista e comunista. "Rinnegato" equivale a traditore; peccato che ci si rivolgesse a chi aveva appena votato la fiducia al Governo dichiarando lealtà al programma elettorale! Merita precisare che quando i 35 deputati così pesantemente apostrofati sono stati eletti, il Popolo della Libertà non esisteva ancora ed in gran parte essi vennero indicati direttamente da Fini all'interno delle liste, e da lui dunque sostanzialmente nominati in Parlamento in virtù delle caratteristiche dell'attuale legge elettorale. Altri si sono riconosciuti in quella destra moderna di libertà e di legalità, di diritti e di responsabilità che Fini ha cercato di rappresentare all'interno del Popolo della Libertà prima di essere di fatto espulso. Credo che la libertà di pensiero, nel rispetto del programma elettorale, non sia ancora vietata in Italia. Curiosa è poi la concezione patrimoniale delle cariche pubbliche che è riecheggiata in quest'Aula. La Presidenza della Camera, nell'intervento qui in discussione, diventa una graziosa e generosa elargizione del Presidente del Consiglio. Questo concetto riporta indietro di 200 anni l'orologio della storia, quando le cariche erano frutto della benevolenza di un principe. Ho lasciato per ultimo il riferimento più sgradevole, lo sprezzante richiamo al copricapo ebraico che Fini sarebbe reo di aver indossato come gesto di omaggio alle vittime della Shoah. Su questi argomenti non è lecito scherzare, com'è inaccettabile definire traditore chi ha condannato la brutalità delle leggi razziali (perché questo è il tradimento che viene rinfacciato all'onorevole Anche in questa denuncia di una pagina ignobile che ha disonorato la storia europea, io sto con Fini, noi stiamo con Fini, come stiamo dalla parte di quella bambina di nove anni, Liliana Segre, il cui racconto mi colpì in modo particolare,

Appena arrivati nel campo di concentramento, venne strappata a suo padre, che finirà in un forno crematorio, come vi finirono sua madre ed i suoi nonni. Chi non capisce l'aberrazione morale di tutti coloro che furono responsabili di quei fatti, ha perso la dignità che deve caratterizzare una persona umana, e lo dico con tristezza sincera. Spiace leggere nel Resoconto stenografico che alcuni colleghi abbiano trovato il cattivo gusto di applaudire le farneticazioni dell'intervento che oggi viene discusso. La politica, se non ritrova rispetto, umanità, saggezza ed equilibrio rischia di portare questo Paese in un baratro oscuro. Non dobbiamo permetterlo; tutti insieme dobbiamo

che il senatore Ciarrapico fece riferimento alle *kippah*, ossia al copricapo ebraico simbolo del popolo di Israele. Voglio ricordare in quest'Aula che tra il 1938 ed il 1945 molti ebrei furono perseguitati in Italia; voglio ricordare quello che accadde nella cosiddetta Notte dei cristalli; voglio ricordare quello che semina l'intolleranza, la persecuzione degli ebrei durante il nazismo; voglio ricordare le conseguenze delle idee, di quell'ideologia tedesca proclamata da Hitler nel «Mein Kampf*»*. Il regime nazista adottò misure sistematiche contro gli ebrei sin dalla sua ascesa al potere in Germania nel gennaio del 1933. Uno dei primi provvedimenti varati si preoccupava infatti di definire chi doveva essere considerato ebreo: era chiunque risultasse avere tre o quattro nonni osservanti della religione ebraica, indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione alla vita dalla comunità ebraica. Mezzo ebreo era chi aveva due nonni osservanti o era sposato con un'ebrea; chi aveva un solo nonno ebreo veniva designato come meticcio. Dal 1933 al 1939 il Partito nazista, enti governativi, banche ed imprese misero in atto un'azione comune volta ad emarginare gli ebrei della vita economica del Paese. I non ariani vennero licenziati dalla pubblica amministrazione; gli avvocati e i medici ebrei persero i clienti ariani; le ditte di proprietà ebraica furono liquidate o acquisite da non ebrei ad un prezzo molto inferiore al valore reale. Il ricavo ottenuto dal trasferimento delle imprese dagli ebrei ai nuovi proprietari e l'arianizzazione dell'economia furono assoggettate a speciali tasse di proprietà. Gli ebrei impiegati in ditte liquidate o arianizzate persero il lavoro. Mi sono permesso di ricordare un pezzo della storia europea, che deve far riflettere tutti,

«A Prato il maltempo fa strage. Annegano tre donne cinesi. Il sindaco dice no al lutto cittadino». proprio in questi giorni ci sarà la visita dal Primo ministro cinese in Italia. Sappiamo che con quell'economia importante in globalizzazione tutti dobbiamo fare i conti, sappiamo che la mancata rivalutazione del renmimbi procurerà dei danni all'economia occidentale e sappiamo che nell'interdipendenza nell'interdipendenza tutti abbiamo bisogno degli altri e che questa intolleranza porta alla ragione che non ragiona più.

Non voglio nemmeno entrare in una giustificazione con distinguo rispetto agli obiettivi di polemica politica del senatore Ciarrapico, che erano probabilmente altri, come egli stesso ha chiarito,

censurato con immediatezza, senza entrare in distinzioni che pur si potrebbero fare - ma che a nulla varrebbero - per ricondurre quella discussione ad una polemica tutta di politica interna italiana e non certo rivolta ad offendere storia, sofferenze, drammi, religioni, Olocausto e quanto di così drammatico e importante è scolpito nella storia della comunità internazionale, e che il popolo ebraico ha patito in Italia e nel mondo. Il

il presidente Berlusconi è stato estremamente chiaro in sede di replica. Noi credevamo, quindi, che le sue parole fossero sufficienti a scandire le posizioni del Popolo della Libertà.

ben conoscono le intenzioni, le politiche e le posizioni del Popolo della Libertà. Credo che la lettera del senatore Ciarrapico, divulgata e riportata con ampiezza,

dunque, discussioni di altra natura, già affrontate anche in quest'Aula, che riguardano, più che le comunità ebraiche, lo Stato di Israele e la sua politica e gli atteggiamenti equivoci di alcuni settori politici nei confronti di chi vorrebbe distruggere Israele e simbolicamente, attraverso gli annunci di distruzione di quello Stato, minaccia nelle sedi ONU e nelle altre sedi internazionali

del Senato le scuse alla comunità ebraica e a tutti coloro che, in qualsiasi parte d'Italia e del mondo, si siano sentiti giustamente offesi da quelle parole. Lo ribadisco in maniera chiara e netta, senza alcuna difficoltà e con sincerità, perché poi le posizioni politiche di ciascuno di noi sono ben note. Non mi dilungo perché il tempo è limitato. Ricordo, però, al di là del Popolo della Libertà, vicende politiche precedenti. Ho a lungo militato in Alleanza Nazionale, e ricordo che nel congresso di Fiuggi uno dei punti salienti fu proprio l'inserimento nelle tesi fondanti di quel partito di affermazioni

c'è convergenza, c'è una doverosa unanimità, che è un fatto di civiltà e di rispetto dei diritti di ciascuno. Riteniamo anche, signor Presidente, con queste ulteriori parole e con le parole, che sono state ricordate, del presidente Schifani, pronunciate grazie a tutti

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le espressioni del senatore Ciarrapico formulate in quest'Aula nel corso della discussione sulla fiducia sono già state duramente e formalmente censurate, sia dal Presidente del Consiglio dei ministri, come è stato detto, nell'immediatezza del fatto, sia dal Presidente del Senato, che anche giustamente ricordato il suo viaggio ad Auschwitz come segno della sua attenzione e dell'attenzione di tutto il Senato al popolo ebraico e alla tragedia dell'Olocausto. Il senatore Ciarrapico, è già stato detto, ha formulato le sue scuse con una lettera aperta nella quale ha chiarito il suo pensiero e che le sue parole non intendevano in alcun modo offendere gli ebrei, ma avevano come unico fine quello di evidenziare l'incoerenza del cammino politico del Presidente della Camera. Quelle parole, pronunciate in quest'Aula, sono state gravemente sbagliate, inopportune e inoltre inutili, perché non accompagnate da alcuna argomentazione seria, e tendenti quindi solo a screditare l'avversario politico, e proprio perciò per noi del tutto inaccettabili. Ribadiamo senza alcuna esitazione la nostra vicinanza e la nostra amicizia con il popolo ebraico e con la comunità ebraica. L'azione di questo Governo è sempre stata attenta alle esigenze della comunità ebraica. Intendiamo quindi stigmatizzare quelle parole, ma permetteteci di dire che ci piacerebbe che analoga reazione di sdegno ci fosse anche in occasione di interventi nelle Aule parlamentari che spesso offendono gravemente il prestigio delle istituzioni di governo. Mi riferisco, colleghi, a quell'epiteto pronunciato dall'onorevole Antonio Di Pietro nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,

e la carica di aggressività manifestata da quelle parole dovrebbe essere condannata fermamente da tutti. Ci saremmo aspettati una reazione sdegnata da parte di tutti: magari non una discussione parlamentare come stamattina, ma almeno una reazione sdegnata. Nessuno Nessuno ha licenza di offendere e di insultare alcuno, sia che si chiami Ciarrapico, sia che si chiami Antonio Di Pietro. Non si può usare, colleghi, un doppio peso basato sulla convenienza politica, per cui se le parole sono pronunciate contro Silvio Berlusconi allora sono espressione di un legittimo diritto di critica politica, nell'ambito della dialettica democratica, mentre se sono pronunciate contro Gianfranco Fini per criticarne i comportamenti politici, allora sono parole inaccettabili, lesive del prestigio delle istituzioni. Il presidente Schifani ha rimarcato giustamente anche in questa occasione che la legittima dialettica democratica non deve degradare in scontro conflittuale fine a se stesso. Abbassiamo tutti i toni, evitiamo le offese a chiunque siano dirette e lasciamo in queste Aule spazio al vero dibattito sui problemi del Paese e alla vera critica politica.

Presidente, intervengo solo per rilevare una nota che a me pare importante: questo dibattito si svolge nell'assenza del senatore Ciarrapico. Ho sentito molte parole, e quasi tutte largamente condivisibili. Però, ho imparato che nella vita contano i gesti, ed il gesto di oggi è di assenza. Ci tengo a ribadire che dal mio punto di vista le scuse

già nei giorni scorsi il presidente Schifani, rispondendo anche alla comunità ebraica, ha stigmatizzato le parole del senatore Ciarrapico.

tutti dovremmo avere più rispetto e abbassare i toni. Tuttavia, qui non si sta discutendo di una critica pesante che qualcuno ha rivolto al Presidente del Consiglio, o della maggiore tutela nei confronti del Presidente della Camera: qui si sta discutendo di un'altra cosa.

evidenziare quello che si ritiene un tradimento, un presunto tradimento politico, un simbolo della religione del popolo ebraico è qualcosa di diverso e di estremamente più grave, su cui il Senato stamattina mi sembra si sia trovato d'accordo. L'Italia e l'Europa hanno gravissime responsabilità nei confronti delle sofferenze degli ebrei e dell'Olocausto: questo è un punto che non si può confondere con la normale, ed anche più bassa, dialettica politica, perché il nostro Paese con le leggi razziali e razziste ha segnato uno dei momenti di vergogna anche della nostra storia. Anche questo oggi è un patrimonio comune, il rispetto, la difesa del popolo ebraico, il diritto alla sicurezza del popolo ebraico nello Stato d'Israele, al di là delle nostre collocazioni, devono rappresentare una questione irrinunciabile, da non confondere - ripeto - con altri aspetti.

il sindaco di Prato ha comunque deciso che ci sia un minuto di silenzio nella riunione del Consiglio comunale, e che la bandiera del Comune sia a mezz'asta. Quindi, si può ritenere questa decisione adeguata o meno, ma non mi pare che sia giusto dire che vi è stato un tapparsi occhi ed orecchi di fronte ad una tragedia che comunque ha riguardato quella città.

il disegno di legge n. 2038, esaminato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, è adesso all'esame del Senato. Ricordo che il testo fu approvato dalla Camera dei deputati da una larghissima maggioranza, 354 voti a favore su 396 presenti. Esso peraltro è il risultato di una unificazione di diverse proposte di legge presentate da tutti i Gruppi parlamentari. Le diverse proposte presentavano contenuti pressoché identici e conseguentemente l'esame alla Camera dei deputati, dapprima presso la Commissione giustizia e successivamente in Assemblea, ha prodotto un testo che, mantenendo ferme le finalità di ciascuna proposta, prevede nei due articoli di cui si compone il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione, espresso in modo chiaro ed inequivoco. In base alla normativa vigente, possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivono abitualmente - anche in parte - con i proventi di attività delittuose; sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisico-morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Come sostenuto in più occasioni alla Camera dei deputati, l'approvazione delle disposizioni è finalizzata a superare la contraddizione in base alla quale ad un sorvegliato speciale è inibita la legittimazione elettorale attiva e passiva, ma non è vietata la partecipazione attiva alle campagne elettorali. Come hanno dimostrato numerose vicende giudiziarie di criminalità mafiosa e come hanno confermato le conclusioni dell'attività di indagine compiuta, nel corso degli anni, dalle diverse Commissioni parlamentari antimafia, il momento principale in cui si realizza la collusione tra criminalità organizzata e politica la fase elettorale, durante la quale può aver luogo l'offerta di voti in cambio di futuri favori da parte di persone soggette a sorveglianza speciale. Lo stesso articolo 416-*ter* del codice penale, che punisce il cosiddetto voto di scambio, si è dimostrato di per sé non sufficientemente idoneo a scongiurare tali rischi collusivi: la fattispecie opera, infatti, solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore. Di qui la necessità di inserire, all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, («Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»), due commi, con i quali si prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni al sorvegliato speciale che svolga attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. La stessa pena si applica anche al candidato che si serva di tale propaganda. Un aspetto discusso, sia alla Camera dei deputati che in Commissione, è quello concernente l'espresso riferimento operato dalla norma alle sole ipotesi di attività di propaganda elettorale prevista dalla legge 4 aprile 1956, n. 212. L'Italia dei Valori ha presentato un emendamento anche in Assemblea, volto a sopprimere il riferimento alla citata legge, esprimendo la preoccupazione che possano essere escluse dalla fattispecie penale modalità di campagna elettorale non espressamente disciplinate da quella legge. La Camera dei deputati ha tuttavia ritenuto di introdurre un espresso richiamo alle norme del 1956, allo scopo di tipizzare la condotta criminosa, limitandola alle ipotesi di campagna elettorale diretta, tra cui rientrano l'affissione dei manifesti, il volantinaggio, i comizi e tutto ciò che viene disciplinato dalla legge. La *ratio* di tale limitazione può probabilmente rinvenirsi nella volontà di scongiurare il rischio di un'eccessiva discrezionalità in sede di individuazione della condotta criminosa, con il conseguente pericolo di improprie strumentalizzazioni a danno di candidati. D'altra parte, solo una norma così strutturata appare corrispondente al principio costituzionale della determinatezza della fattispecie penale. Ai sensi del nuovo articolo 5-*bis*.2, il coinvolgimento del candidato dovrà essere provato attraverso elementi certi ed obiettivi,

e, nello stesso tempo, richieda consapevolmente al medesimo soggetto la propaganda elettorale, se ne avvalga concretamente o comunque ne usufruisca. La condotta punibile del candidato, pertanto, è integrata quando questi inequivocabilmente sia a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e vi sia una richiesta di detta attività. Rafforza tale fattispecie, poi, la previsione che l'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse rispetto alle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Il coinvolgimento, quindi, deve fondarsi su elementi certi ed obiettivi e non, ad esempio, sul semplice ritrovamento di un volantino di sostegno elettorale nell'abitazione del pregiudicato. Quanto infine alle conseguenze in caso di condanna, occorre sottolineare l'equiparazione prevista tra la condanna e la pena patteggiata. Ciò al fine di evitare che il patteggiamento possa essere una via per eludere le importanti conseguenze previste per la condanna stessa. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva: a tal fine, la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo competente dell'ente di appartenenza per l'adozione degli atti conseguenti. Alla misura interdittiva consegue l'ineleggibilità del soggetto per la stessa durata della pena detentiva comminata, e la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici. Per queste ragioni ritengo di dover sottoporre all'attenzione dell'Aula la necessità dell'approvazione del provvedimento nello stesso testo in cui è stato approvato dell'altro ramo del Parlamento, perché possa entrare immediatamente in vigore facendo, ancora una volta, chiarezza e pulizia sui rapporti tra mafia e politica.

la ringrazio; occuperò anche meno del tempo che mi è concesso. Condividiamo questo disegno di legge, che introduce una fattispecie di reato che va a coprire le attività di propaganda elettorale da parte di un sorvegliato speciale. Indubbiamente, la previsione di inibire un ruolo attivo nel corso delle elezioni a soggetti che per legge non hanno l'elettorato, né passivo, né attivo, colma un possibile aggiramento dello scopo che aveva la normativa attuale, così estendendo anche alle attività di propaganda, ovviamente con le garanzie richieste in ordine alla certezza e alla consapevolezza del candidato, il divieto di quelle condotte che, specie in alcune realtà, potrebbero costituire spesso la storia giudiziaria del nostro Paese lo ha dimostrato - delle forme di condizionamento del voto da parte di soggetti che, proprio per lo stato giuridico di cui sono portatori, dovrebbero essere neutralizzati in un momento così importante della vita democratica del Paese. Siamo quindi d'accordo; le nostre perplessità e i nostri emendamenti tendevano a superare quegli errori tecnici che questo testo contiene. Il riferimento alla propaganda elettorale, così come definita dalla legge n. 212 del 1956, ci appariva riduttivo, dal momento che la legge in questione fa esclusivo riferimento al al volantinaggio, all'affissione di manifesti e al divieto di propaganda elettorale nei giorni di silenzio imposti dalla legge. Ci sono altre fonti normative che individuano il concetto di propaganda elettorale, ad esempio la legge n. 28 del 2000, che riguarda la stampa e la trasmissione radiotelevisiva, forme di propaganda elettorale molto più invasive e attuali rispetto al volantinaggio e all'affissione di manifesti; sicché ci pareva che il richiamo contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge al divieto di propaganda elettorale previsto dalla legge n. 212 del 1956, ossia l'affissione di manifesti e il volantinaggio, fosse riduttivo rispetto all'obiettivo che la legge vuole perseguire. la nostra proposta suggeriamo di omettere il riferimento alla legge n. 212 del 1956, non essendo l'unica legge che definisce la propaganda elettorale,

dobbiamo licenziare questo disegno di legge, perché tutti lo condividiamo, ma tecnicamente rappresenta un passo indietro rispetto a ciò che il nostro sistema già prevede. Il nostro sistema, all'articolo 28 e 29 del codice penale, prevede che, se le pene per i delitti sono superiori a cinque anni, l'interdizione è perpetua; se le pene per delitti sono comprese tra i tre e i cinque, anni l'interdizione è di cinque anni; non è invece prevista interdizione per le pene inferiori ai tre anni.

viene condannato ad una pena di cinque anni in virtù di questa legge l'interdizione sarà di cinque anni, mentre per il nostro codice l'interdizione sarebbe perpetua. si viene condannati ad una pena di tre anni, in virtù di questo disegno di legge l'interdizione è pari a tre anni, mentre il nostro codice prevede che sia pari a cinque anni. Ritengo invece positiva l'interdizione, che il nostro attuale sistema non contempla, per le pene inferiori ai tre anni. Di fronte a questo errore tecnico che indebolisce il sistema delle interdizioni previsto dal nostro codice, nel momento in cui avvertiamo la necessità di intervenire con questo disegno di legge disciplinando la materia e introducendo questo tipo di reato, per quale motivo dovremmo essere censurabili avendo introdotto un sistema più debole di quello previsto

In Commissione abbiamo ritirato gli emendamenti riservandoci di presentarli in Aula. Vogliamo lanciare un messaggio al Paese? Possiamo approvare il provvedimento così com'è, ma contiene

Proprio nel momento in cui avvertiamo l'esigenza di introdurre questo reato indeboliamo la normativa sanzionatoria, con una profonda contraddizione in termini. Qualcuno ci criticherà per il nostro per il nostro errore tecnico, per avere infranto il sistema previsto dal codice penale essendo scontato che questa legge, essendo speciale, prevale sulla norma generale e ordinaria del codice penale. Ci prenderemo le critiche di qualche osservatore attento; ci diranno che non siamo dei buoni legislatori. Vogliamo pagare questo costo? Paghiamolo, posso rinunziare agli emendamenti; però forse una correzione con un altro passaggio veloce in Aula esclusivamente limitato a questo punto consentirebbe di fare un prodotto compiuto ed in linea con il nostro sistema: raggiungeremmo il risultato, sia pure con un ritardo di due o tre settimane, tre settimane, elaborando un prodotto giuridicamente corretto. Mi affido alla sensibilità dei colleghi;

da tanti anni fa. Nel momento in cui ci arriviamo, arriviamoci bene. Affido alla sensibilità degli altri Gruppi se coltivare o meno questi nostri emendamenti, che metto a disposizione

Signor Presidente, colleghi senatori, innanzitutto prendiamo favorevolmente atto delle considerazioni del senatore Li Gotti e e attendiamo la risposta del Sottosegretario per cercare di capire meglio la questione. Il testo in esame offre l'opportunità di colmare un'annosa lacuna in materia di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella sfera politica. In tale ambito sarebbe stato lecito attendersi un intervento ben più sollecito da parte del legislatore. Si tratta di un'aspettativa, al contrario, lungamente insoddisfatta, tanto che agli elementi contigui alle organizzazioni criminali, pur sottoposti a misure di prevenzione per circoscriverne la pericolosità sociale, è stato possibile sostenere attivamente candidature elettorali compiacenti, inoculando così nei gangli vitali dello Stato il germe del malaffare. Rallegriamoci, dunque, nel constatare la maturata consapevolezza politica che, oggi, guadagna il battimano a chi afferma la necessità di prevenire il rischio e l'onta di poco raccomandabili intrusioni. Rallegriamocene, colleghi senatori, come di una conquista sofferta, perché, a parte i tempi lunghi dell'attesa, vi fu chi sollevò la questione e certo non conobbe gli applausi tributati a quanti intervengono in quest'Aula sull'argomento. Al contrario, poteva capitare che un sindaco desse comunicazione al suo partito circa il via vai di noti camorristi tra i seggi elettorali e che per tutta risposta venisse trattato da anima bella, che gli si ridesse in faccia, che lo si inducesse a togliere il disturbo. Guardate che accadeva soltanto cinque anni fa a Ersilia Salvato, già primo cittadino di Castellamare di Stabia e senatrice dei Democratici di Sinistra, costretta a lasciare il partito dei DS di fronte al muro di disinteresse e ostilità che, come lei stessa rivelò agli organi di informazione, fece seguito alla sua, inascoltata, denuncia di attivismo camorrista nella campagna elettorale. D'altro canto, al profluvio di fiato e inchiostro sparso da politici e opinionisti nel paventare le penetrazioni mafiose nella cosa pubblica, la compravendita dei consensi, la manipolazione del voto, si è accompagnato il regime "antimafia", imposto ai cosiddetti sorvegliati speciali dalla legge n. 575 del 1965, che non andava oltre la preclusione di accedere o mantenere licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni, appalti ed erogazioni da parte dello Stato. Finalmente le modifiche alla suddetta normativa, ora opportunamente integrata dal divieto dello svolgimento di propaganda pro o contro candidati di qualsiasi competizione elettorale, prendono in considerazione il momento elettorale, cioè la più alta espressione della vita democratica, come un bene bisognoso di particolare tutela dalla minaccia mafiosa. E, innegabilmente, il disegno di legge in discussione appare adeguato allo scopo, in virtù della previsione delle severe pene detentive per i trasgressori, puniti con la reclusione sino a cinque Alla medesima sanzione soggiace il candidato che si avvalga del sostegno illecito: circostanza ben ponderata nella definizione normativa, come dimostra la richiesta che l'ipotesi di reato venga accertata tramite l'acquisizione di prove ulteriori in aggiunta alla semplice chiamata in reità da parte del sorvegliato speciale. Basterà tale accorgimento, caro Presidente, per scongiurare l'eventualità che la norma si trasformi in un'arma a doppio taglio? Basterà il previsto circoscritto ridimensionamento del pentitismo a togliere dalle mani delle organizzazioni criminali lo strumento della calunnia in sede giudiziaria? Basterà questo per allontanare la spada di Damocle dal capo di politici scomodi o refrattari agli interessi mafiosi? Ce lo auguriamo vivamente, confidando in un operato della magistratura necessariamente prudenziale, considerato il pericolo che un impiego garibaldino della presente normativa comporterebbe per la giustizia e la stessa democrazia. Tale aspetto di criticità, d'altronde, non scalfisce l'alto valore, anche simbolico, intrinseco nel provvedimento in esame. Finalmente la legge proclama, anzi ingiunge, che mai più venga tollerato alcun commercio tra lo Stato e l'anti-Stato, mai più la commistione tra il delegato dei cittadini e il manutengolo del malaffare, mai più l'equivoco tra l'interesse generale e l'iniquità prevaricatrice.

Signor Presidente, ci troviamo in un periodo, a mio avviso, in cui bisogna prestare una diversa e particolare attenzione al tema della criminalità organizzata, che rifletta il dato che questa nostra società abbia preso coscienza e consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata non si fa più soltanto con convegni, con dichiarazioni o con enunciazioni di principio, né tanto meno esclusivamente con il professionismo dell'antimafia. Allora, questo aspetto e questo dato ci riportano pienamente ad un clima nuovo, che noi vogliamo creare all'interno delle realtà dei territori per isolare sempre più la criminalità organizzata, ma soprattutto per togliere la possibilità a chi pensa, pur essendo criminale, di poter gestire campagne elettorali e quindi avere sempre più un rilievo, un'attenzione e un ruolo sociale molto forti. Qui non è in gioco il contrasto o la lotta a una determinata cosca, ma sono in gioco la cultura, la civiltà, la democrazia e la libertà all'interno del nostro Paese. È bene sottolineare che il problema delle cointeressenze tra politica e mafie non riguarda soltanto il Mezzogiorno, tuttavia in alcune Regioni, soprattutto del Mezzogiorno, il peso e la pervasività delle mafie e delle organizzazioni criminali rende assai difficile l'esercizio della rappresentanza e il lavoro delle istituzioni. Questo disegno di legge nasce dalle iniziative di molti parlamentari del Mezzogiorno, perché sono quelli che vivono in queste Regioni e che conoscono quanto importante e decisiva per lo sviluppo di questi territori sia l'attività di contrasto alle mafie, a cominciare dai comportamenti che riguardano la politica. Sono state avanzate diverse osservazioni sul fatto che questa norma potrebbe prestarsi a un uso strumentale. Dov'è questo uso strumentale, se si prevede che la responsabilità del candidato debba essere accertata con sentenza definitiva? Dov'è questo uso strumentale, se nel testo si prevede che il candidato debba avere consapevolmente richiesto lo svolgimento di campagna elettorale ai mafiosi? Riteniamo che non ci sia alcuna lesione dei diritti civili e della libertà. Anzi, ci stupiamo che qualcuno ne parli, perché gli effetti di questo provvedimento si producono solo in presenza di una sentenza definitiva. Allora, cosa dire della legge sullo scioglimento dei consigli comunali che colpisce tutti i consiglieri, sia quelli che hanno avuto rapporti con la mafia, sia quelli che non hanno avuto tali rapporti? Questo provvedimento almeno colpisce quelli che deliberatamente hanno richiesto ai mafiosi un sostegno in campagna elettorale. Non si tratta, quindi, di dividersi tra garantisti e giustizialisti, ma neanche di nascondersi dietro un garantismo di facciata e di nascondere dietro a ciò un eccesso di zelo nella tutela delle garanzie della politica e di quanti fanno politica. Se si trattasse di scegliere tra questo garantismo di facciata, questo eccesso di zelo nella difesa e nella tutela delle garanzie dei politici e i diritti e le libertà dei cittadini che, soprattutto in alcune parti del Paese, vivono l'assenza di libertà e la negazione dei diritti a causa della presenza assillante della mafia, allora non avremmo alcuna difficoltà a scegliere tra le due cose, ovvero l'approvazione di questo provvedimento, ritenendo questo testo necessario. Tutti sappiamo che i partiti, in prossimità di ogni campagna elettorale, licenziano dei codici etici che dovrebbero schermare la politica da ogni complicità con la 'ndrangheta, la mafia e la camorra. Tutti però verifichiamo, dopo ogni campagna elettorale, quanto questi codici etici non siano stati sufficienti a raggiungere l'obiettivo. La mafia, la 'ndrangheta e la camorra spesso, quando devono scegliere chi sostenere alle elezioni, facendo leva anche sulla competizione che le elezioni stesse generano, sostengono quelli che sono capaci di passare indenni il vaglio dei codici etici dei partiti. Concludo dicendo che è un testo che ha il pregio di rendere inutilizzabili i voti della mafia. In campagna elettorale spesso si ascolta quanti dicono che tutti i voti sono uguali e che i voti non hanno odore. Spesso questo diventa un alibi nel ricercare voti in qualsiasi contesto. Ebbene, con questa legge si dice che i voti ottenuti dalla mafia sono inutili per chi è impegnato in campagna elettorale. Questo è il pregio del testo che oggi approviamo: quello di dimostrare che c'è una politica che non vuole più ritenere che tutti i voti siano legittimi, ma che ci sono alcuni voti che uccidono la speranza di certi territori. Ed ancora, a quanti lamentano che in questo testo ci sarebbe la possibilità di una lesione dei diritti e delle libertà, vorrei far presente che l'esercizio delle elezioni, attraverso le candidature e i candidati, è innanzitutto un esercizio utile ad affermare i diritti e le libertà dei cittadini che, soprattutto in alcune parti del Paese, vorrebbero una politica coraggiosa, al punto da rinunciare a un eccesso di zelo nella difesa delle proprie garanzie, se a questa rinuncia può corrispondere una norma capace di aiutare anche i partiti e i politici a fare in modo che non si faccia di tutta l'erba un fascio e che anche nelle Regioni del Mezzogiorno si possa dire che c'è una politica che rifiuta certi voti, perché non è vero che certi voti non hanno odore.

pratica, il cuore del provvedimento, il nucleo fondamentale del testo è l'introduzione, nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto di svolgere, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, le attività di propaganda elettorale, rispetto a qualsiasi tipo di competizione elettorale, a favore o contro candidati o simboli. Questo è il cuore del provvedimento normativo e un'incongruenza forte di tipo legislativo. Infatti, secondo la normativa finora vigente, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

che abitualmente commettono reati di diverso tipo, ma naturalmente la preoccupazione e la casistica più ampia riguardano le persone che, in modo singolo o associato,

ma non impedisca loro di svolgere propaganda elettorale nei diversi contesti. È già stato rilevato come questa legge rappresenti l'acquisizione all'interno del testo di un punto di vista anche culturale e politico su come si combatte la malavita organizzata e di come si possa colpire quel rapporto tra politica e malavita organizzata che la legge attuale - mi riferisco alla questione già posta da altri colleghi del voto di scambio - riconduce solo

di combattere questo fenomeno poiché è nel momento della campagna elettorale che si crea una collusione tra malavita organizzata e alcuni esponenti della politica, che si traduce in campagna a favore o intimidazioni anche nei confronti di altri candidati o di elettori. Da ciò scaturisce un fenomeno davvero inquinante

emersi in quest'ultimo periodo nella Regione in cui vivo, non riguarda solamente il Mezzogiorno. Si tratta quindi di una misura molto opportuna perché - come ho detto - è appunto nella fase elettorale che si stringono quei rapporti sulla base dei quali esponenti della criminalità organizzata offrono voti in favore di candidati, in cambio di favori futuri che possono ottenere - e spesso ottengono, purtroppo - negli affari pubblici, in particolare negli appalti.

Grazie

di essere preda della rassegnazione, della disaffezione rispetto alla politica e dell'idea che nulla mai possa cambiare. Diamo un segnale

n. 575 del 1965, non contemplava infatti l'irrogazione di una misura interdittiva all'esercizio dei diritti politici nei confronti delle persone che fossero state assoggettate ad una misura antimafia quale, appunto, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Potevamo e possiamo dire che c'era una carenza assiologica di copertura delle misure di prevenzione proprio su questo delicatissimo settore, che involge le relazioni tra le istituzioni e l'esercizio dei diritti politici. Possiamo anche aggiungere, signora Presidente e onorevoli colleghi,

particolare, accanto alle classiche disposizioni che prevedono la compressione del diritto di elettorato passivo e attivo nei casi

di nessun candidato alle elezioni politiche, né a quelle amministrative. Signora Presidente, onorevoli colleghi, al di là delle affermazioni che sono state qui ripetute da molti colleghi, credo che questa sia una disposizione di grande spessore e chiarezza normativa e sia, se mi è consentito, anche una norma che va ad irrobustire il tessuto e gli anticorpi che possono rendere le istituzioni democratiche sempre più forti e impermeabili alle infiltrazioni criminali e, in particolare, a quelle proprie di organizzazioni mafiose o criminali. In questo contesto, in questa cornice istituzionale, la disposizione che è stata portata all'approvazione del Parlamento credo che possa naturalmente indirizzare anche il circuito istituzionale ad un comportamento etico che sicuramente, anche sulla base delle disposizioni del codice etico che la Commissione parlamentare antimafia ha elaborato,

Se avessimo avuto un po' di tempo non mi sarebbe dispiaciuto presentare modifiche che potessero intervenire anche sul sistema sanzionatorio. Penso, infatti, che questa fattispecie incriminatrice dovrebbe essere punita con sanzioni che possano permettere l'arresto in flagranza di reato. Naturalmente il sistema sanzionatorio di questi illeciti deve essere ben parametrato con il principio di ragionevolezza delle leggi di cui all'articolo 3 della Costituzione e anche

che i criminali, e in particolare coloro i quali sono sospettati di appartenere a organizzazioni mafiose, non solo non godono di alcun diritto politico, ma non possono neppure interferire in modo indiretto sulle campagne elettorali e sui processi di selezione della classe dirigente del nostro Paese. La ringrazio, signora Presidente. Ringrazio anche il relatore, presidente Vizzini, per la celerità e la competenza, ma soprattutto per la capacità e la caparbietà con cui ha sostenuto questo provvedimento. Grazie di cuore, signora

il disegno di legge in materia di svolgimento della propaganda elettorale da parte di persone soggette a misure di prevenzione giunge all'esame dell'Assemblea dopo approfondite discussioni presso la Camera dei deputati, dove ha preso forma

del provvedimento stesso e che il Governo si dichiara disponibile ad accogliere. Verrà così colmato un vuoto normativo e si ostacoleranno la disponibilità del malavitoso e l'affidamento a questi del candidato nella fase elettorale dove maggiormente si registra in modo visibile la stretta collusione tra la politica e la criminalità organizzata. Viene introdotto il divieto di svolgimento della propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione in forza di provvedimenti definitivi, L'intento è quello di recidere il rapporto tra la politica inquinata, le zone grigie e le criminalità organizzate: un rapporto nefasto, particolarmente radicato in alcune zone del Paese, contro cui il Governo e il Ministero dell'interno sono concretamente impegnati. Per tali ragioni, viene anche sanzionata la condotta del candidato che, per lo svolgimento della propria propaganda elettorale, si rivolge, cercandone l'aiuto, a persone sottoposte a misure di prevenzione. L'approvazione del disegno di legge consentirà, allora, di ottenere il duplice effetto di rendere molto complesso al malavitoso e molto rischioso al candidato l'appoggio elettorale, ad iniziare dall'esibizione, che è un tipico atto intimidatorio e coercitivo nei confronti del corpo elettorale. Si combatte anche in questo modo una grave distorsione della rappresentanza politica e, dunque, della democrazia nel nostro Paese, nonché si contribuisce a togliere spazio ai sistemi criminali e ai comportamenti equivoci. Una menzione meritano l'impegno della società civile e la passione per la legalità di numerosi studiosi, tra cui quelli del Centro studi Lazzati di Lamezia Terme, che da lungo tempo auspicano le misure in votazione.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

4 aprile 1956, n. 212». In questo modo, il riferimento normativo renderebbe applicabile a tutte le forme di propaganda la norma che si intende introdurre.

La 1a Commissione permanente, come il relatore con la consueta onestà intellettuale ha detto, ha convenuto sul fatto che occorreva dare un segnale che potesse essere tempestivo. Infatti, con

Sono emendamenti che in linea di massima condividiamo e corrispondono ad esigenze effettive che potranno essere riconsiderate

ci sono segni preoccupanti di un forte, crescente interesse delle organizzazioni criminali nei confronti della politica, con una serie di attentati anche ai danni di amministratori locali e sindaci. Riteniamo preferibile dare un segnale forte ed unitario: il Parlamento approvi oggi in via definitiva il disegno di legge

la nostra forte richiesta, se lo valuteranno opportuno, di trasformarli in un ordine del giorno. Tra l'altro, signora Presidente, uno degli emendamenti ha un carattere essenzialmente interpretativo,

numerosi territori, e cioè che molti sorvegliati speciali nel momento *clou* della campagna elettorale sono presenti ed esercitano la loro forza e il loro valore simbolico mettendo a servizio di candidati compiacenti la loro capacità di raccogliere voti e di pressare cittadini onesti in tale direzione. Sono anche d'accordo a che questo provvedimento sia approvato qui oggi, al Senato, ma anch'io voglio sottolineare che forse alla Camera

Un aspetto ha bisogno di un ritorno legislativo: quello relativo all'interdizione dai pubblici uffici, perché è vero che c'è una incongruenza e bisogna fare in modo che questa sia superata con un intervento legislativo, e quindi con una correzione normativa, in modo tale da portare tale da portare in equilibrio l'interdizione prevista in questo caso nei confronti del sorvegliato e del candidato compiacente

tentare di dare un'interpretazione estensiva autorevole da parte del Parlamento, ma c'è anche un'altra incongruenza che forse alla Camera

mentre per tutte le altre utilità, che sempre più sono il canale intorno a cui si salda il rapporto politico-mafioso in campagna elettorale, non è prevista alcuna sanzione.

nonostante avessimo alcune perplessità di merito, su una questione impropriamente definita Piano straordinario antimafia perché da parte del ministro Maroni ci era stata data garanzia che alla ripresa dei lavori avremmo avuto uno strumento normativo per intervenire e colmare i buchi che c'erano in quel provvedimento, e che adesso registriamo anche

perché abbiamo bisogno di fare una buona antimafia, e una buona antimafia si fa quando le norme sono prive di così enormi contraddizioni e sono in grado realmente di essere efficaci di essere efficaci al momento dell'attuazione. Ecco perché ho voluto sottolineare questi punti: perché vi faremo sentire la nostra voce in Parlamento e segnaleremo le contraddizioni, tutte le volte che si presenteranno. Vi invitiamo sul serio

limitandoci solo a dei proclami. C'è bisogno che il Parlamento faccia scelte che mai nella storia del nostro Paese ha fatto. Ed è possibile farlo oggi, perché ci sono norme

5-*bis*.2. Vedete, trattandosi di norma penale, e quindi di stretta interpretazione, per la quale - come sappiamo - è vietata l'interpretazione analogica, si punisce gravemente con la reclusione da uno a cinque anni un soggetto, in quella particolare condizione di essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quando svolga l'attività di propaganda in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale; invece non è possibile applicare la stessa norma nei confronti di quei soggetti che svolgano eventualmente attività di propaganda in favore di forze politiche e di partiti politici o di soggetti politici. Non c'è nessun interprete che voglia essere attento ai parametri ermeneutici del diritto penale che possa poi stabilire la punibilità di questo comportamento se il soggetto non fa propaganda a favore di uno o più candidati, come prevede la norma, ma a favore di una forza politica, quale che essa sia. Questo è il limite. Devo esprimere questa perplessità, perché non posso farne a meno. Poi voterò il

l'opportunità di approvare oggi il provvedimento e farlo diventare legge possa suggerire a tutti l'idea di una trasformazione degli emendamenti in un ordine del giorno che riassuma le osservazioni del collega Li Gotti e che può diventare strumento da riportare presto all'esame del Parlamento, anche in attesa di provvedimenti che il Governo aveva annunciato e che potrebbero consentire che ciò accada. Lo dico anche in riferimento al metodo che fu adottato - come ricordava il collega Lumia - in occasione dell'approvazione del disegno di legge del Governo che stabiliva la redazione del codice antimafia e una serie di altre misure.

contiene delle lacune che è necessario eliminare, non escluso anche l'ulteriore limite che è stato indicato dal senatore Longo, ossia il fatto che l'impostazione di questa legge vieta la propaganda elettorale a favore o contro il candidato, ma non a favore o contro il soggetto politico o il partito. Anche questo è indubbiamente un suggerimento che potremmo recepire, il Senato può portare il suo concreto contributo a questa legge, così come essa merita. Raccolgo quindi la sollecitazione: votiamo all'unanimità il provvedimento in esame, ma il Senato ha la competenza e l'autorevolezza per intervenire e migliorare questo testo legislativo.

con riferimento alle questioni che sono state sollevate. Ad esempio, il rinvio alla legge n. 212 del 1956 può essere specificato nell'ordine del giorno, e questo, verosimilmente, potrebbe anche andare incontro ai dubbi sollevati, chiarendo che si fa riferimento a

Presidente, già il collega Bianco nel suo intervento aveva esposto gli stessi suggerimenti e gli stessi intendimenti che il collega D'Alia ha

come è già stato ricordato sono molti gli anni e le legislature in cui si è provato ad affrontare i temi proposti con questo provvedimento. Io stesso avevo presentato già nella scorsa legislatura un disegno di legge sull'argomento. È da tempo che in particolare i parlamentari del Sud, anche grazie alle sollecitazioni del Centro studi Lazzati e del suo presidente, dottor Romano De Grazia, provano ad introdurre un ragionamento semplice per contribuire a stroncare un intreccio perverso. Tuttavia le resistenze sono state tante e tali che solo in questo ultimo periodo sembra concretizzarsi la possibilità di approvare tali provvedimenti. Resistenze di merito e di principio hanno ostacolato tali decisioni negli anni passati. Ed anche per questo forse vale la pena soffermarsi un attimo di più in quest'Aula sul tema. Il ragionamento proposto è che non si comprende bene la logica secondo la quale ad un sorvegliato speciale viene sottratto l'elettorato attivo e passivo mentre resta libero di svolgere attività elettorale a favore di candidati o di simboli o di partiti, che spesso sono consapevoli di rivolgersi a personaggi in grado di influenzare il voto elettorale. Parliamo di sorvegliati speciali: di soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi, che vivono con i proventi di attività delittuose, che sono dediti alla commissione di reati e spesso indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Per tali soggetti si propone il divieto di propaganda elettorale, mentre si propone una sanzione per quel candidato che si rivolge coscientemente al sorvegliato speciale nella richiesta di sostegno elettorale. Quello che, in buona sostanza, questo disegno di legge si propone è di spezzare l'intreccio perverso a cui accennavo poc'anzi. Si tratta di rendere più complicata, e sanzionabile, la possibilità che si realizzi un legame tra soggetti e organizzazioni criminali e candidati ed organizzazioni politiche. Si prova cioè a colpire i criminali in una parte del loro patrimonio: nell'influenza che, attraverso metodi coercitivi o meno, esercitano nelle comunità in cui sono insediati. Anche perché il fenomeno ha ormai assunto caratterizzazioni che non solo riguardano pezzi della politica, ma arrivano al complesso delle istituzioni. A molte organizzazioni criminali non importa chi si afferma durante le elezioni: anzi, se si ravvisa la possibilità che una parte sia nettamente vincente, è proprio verso quella direzione che si appuntano le maggiori attenzioni per stringere, proprio nella fase elettorale, come mostrano molte indagini e risultanze investigative, veri e propri accordi sui futuri comportamenti e atti da adottare. Oggi - devo dire purtroppo - si sono creati un clima e un'attenzione che forse consentiranno di tradurre in norma l'impegno di tanti che si sono spesi in questa direzione. Dico purtroppo perché, in qualche modo, ci sono voluti episodi come le auto cariche di armi e di esplosivo di esplosivo sul percorso del Presidente della Repubblica, i troppi bazooka ritrovati, gli attentati alla magistratura o alle forze dell'ordine, le intimidazioni agli amministratori, agli imprenditori e ai giornalisti

nella sanità, nella gestione del mercato clandestino dei braccianti agricoli, negli appalti vinti dalle grandi imprese di Stato, sempre troppo pronte a pagare tangenti anche mediante pratiche di subappalto. C'è voluto tutto ciò per operare un salto di qualità dall'antimafia del chiacchiericcio, delle passerelle e dei convegni all'azione convinta del Parlamento e di tutte le istituzioni nel fronteggiare una piaga e un freno allo sviluppo del Sud. Io poi ho un altro motivo per sentirmi soddisfatto: questo questo è un provvedimento fortemente sostenuto dalla classe dirigente politica calabrese. Vedete, la scena della donna e dei parenti che applaudivano il boss mentre la volante della polizia lo portava via ha fatto il giro del mondo. Ha scomodato esperti di sociologia, di antimafia, consulenti tuttologi e perfino illustri antropologi (qualche giornale di qualche forza politica ha fatto scrivere sul tema trattati ad antropologi): tutti ad analizzare il caso Reggio Calabria con un sottofondo particolare: si sussurrava che «nemmeno in Sicilia...». Persino in Sicilia l'opinione pubblica reagiva, mentre a Reggio si applaudivano i boss. Non era affatto vero. Tanto per citarne una, qualche giorno addietro c'è stata una straordinaria manifestazione di piazza contro la 'ndrangheta a cui migliaia e migliaia di calabresi hanno partecipato per sostenere i magistrati e tutti i calabresi onesti e perbene. Peccato sia passato tutto nell'indifferenza dell'opinione pubblica nazionale! Convenienze economiche che sposano precise convenienze politiche ben saldate nelle paure del Nord non trovano né la voglia, né l'onestà per raccontare l'altro Sud: quello che non si arrende e non si piega alla criminalità e alle commistioni tra politica e criminalità. Oggi quel Sud, probabilmente nel silenzio generalizzato dei media nazionali, registra un altro colpo a suo favore: spinge anche il Senato ad approvare questa legge. Forse è un atto più simbolico che effettivo, ma la nostra società si nutre anche di simboli, oltre che di volontà. Per noi questo è un atto importante. Per noi questo è un ottimo giorno. In Calabria, signora Presidente, si rischia di finire come in Sicilia ai tempi di Falcone e Borsellino: il Parlamento, il Governo e tutte le istituzioni devono intervenire immediatamente, prima che dalla strategia della tensione si passi a colpire uomini dello Stato e delle istituzioni. Per questo c'è bisogno che il Parlamento stia accanto alla gente del Sud, per questo c'è bisogno che la Presidenza solleciti i ministri Maroni e Alfano a venire in Aula a riferire sulle questioni che riguardano la Calabria. Per questo noi di Alleanza per l'Italia esprimiamo convintamente un voto a sostegno del provvedimento. onorevoli colleghi, sicuramente il provvedimento che ci apprestiamo a votare, e per il quale il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà un voto decisamente favorevole,

previsto, nell'autoregolamentazione di condotta dei partiti che si presentano alle elezioni, la non candidabilità (sotto forma di autoregolamentazione, di coloro nei cui confronti era stata applicata la misura di prevenzione personale o patrimoniale, ai sensi della legge n. 575 del 1965. Questo è quello che la Commissione antimafia all'unanimità ha approvato. Rimaneva però l'aspetto per cui si sollecitavano le forze politiche a non candidare questi soggetti, ma non era prevista alcuna norma che impedisse agli stessi di svolgere propaganda elettorale, a favore o contro. E la propaganda elettorale di questi soggetti, a favore o contro, non è la normale propaganda elettorale, il che avrebbe potuto far ritenere addirittura incostituzionale una disciplina del genere, perché si tratterebbe di vietare ad un cittadino la possibilità di esprimere e di fare conoscere il proprio orientamento sollecitando l'adesione sulle proprie idee. No, noi stiamo parlando della condizione soggettiva e della particolare «propaganda elettorale» che un soggetto ritenuto pericoloso per la società fa nel momento in cui appoggia un candidato o ostacola una candidatura: sono persone che si avvalgono del loro *status* per condizionare il voto. È, purtroppo, storia della nostra democrazia il fatto che spesso nei pressi dei seggi elettorali vengono avvistate le presenze - e basta la presenza in alcuni casi - di malavitosi con la loro presenza condizionano gli elettori. Almeno con questa legge ci dotiamo di uno strumento: il candidato ora deve sapere che qualora

che siano espressione di volontà non coartate o non condizionate. Il nostro voto è, quindi, favorevole. Poi miglioreremo questo testo nel senso che ho auspicato: adegueremo al diritto comune, alla normativa ordinaria del codice penale, lo estenderemo a tutte le forme di propaganda, prevedremo anche la richiesta indiretta al sorvegliato speciale di far propaganda per un partito, raccoglieremo le sollecitazioni del senatore Longo, che ha parlato di prevedere anche la propaganda a favore e contro un soggetto politico qualunque esso sia, la lista o il partito e non solo il candidato.

Lo votiamo perché vogliamo fare un'altra cosa. Pensare che il soggetto pericoloso si metta a distribuire volantini o ad attaccare manifesti prevedere la punizione soltanto di queste condotte è francamente riduttivo rispetto alla realtà che conosciamo. Leggiamo il testo che stiamo per approvare per ciò che ancora non contiene e per come verrà integrato in futuro, perché per quello che contiene è un po' ridicolo. Ma il nostro voto è favorevole.

credo sia il periodo e il giorno giusto perché il Senato e il Parlamento diano una risposta in termini chiari agli attentati e ai tentativi di attentato che hanno riguardato la procura della Repubblica di Reggio Calabria e i magistrati calabresi, che devono sentire quotidianamente il sostegno di tutto il Parlamento, di tutte le forze politiche e di tutte le istituzioni, perché sono in prima linea nel contrasto ad un'organizzazione che è sempre meno criminale e sempre più terroristica. C'è bisogno dell'unità vera delle forze politiche nel contrasto e nella guerra che deve essere fatta. Questo provvedimento, signora Presidente, si inquadra nell'ambito di quell'attività che insieme, maggioranza e opposizione, stiamo facendo in Parlamento per costruire un sistema di regole che sia quanto più possibile efficiente ed efficace rispetto all'evoluzione del fenomeno criminale. È chiaro, ci sono nel testo alcuni aspetti che possono dare adito a diversità di interpretazione, ma con la buona volontà e il buon senso - ringrazio molto il collega Li Gotti in questo senso - e anche con l'ordine del giorno che tutti insieme abbiamo presentato credo che molte di queste perplessità possano essere superate dall'approvazione di quell'ordine del giorno, che ha natura interpretativa, senza bisogno di tornare ad un nuovo intervento legislativo. Tuttavia, qualora questo fosse necessario, abbiamo approvato prima dell'estate un pacchetto di norme antimafia che prevede anche una serie di deleghe relative alla riorganizzazione del quadro normativo di riferimento e i testi unici riguardante il contrasto alla criminalità organizzata e quindi quei dubbi potrebbero essere affrontati e risolti, anche grazie a questo ordine del giorno, in quel provvedimento. Pertanto, credo che oggi noi - e ringrazio il presidente Vizzini - abbiamo fatto un lavoro buono e giusto, e lo abbiamo fatto nell'interesse soprattutto di quegli operatori della giustizia e della sicurezza che devono sentire ogni giorno il conforto della politica, senza alcun tipo di delegittimazione. Lo abbiamo fatto anche nei confronti di tutto il ceto politico, che da oggi deve sapere che anche l'idea di una contiguità più o meno consapevole con determinati ambienti, con determinate persone è motivo di sanzione penale, perché se non introduciamo questi criteri e queste regole, verosimilmente anche l'*humus* della contiguità nel rapporto tra politica e mafia diventa un elemento destabilizzante. Questo è il senso di questa iniziativa legislativa fortemente voluta da alcuni esponenti della società civile calabrese, e credo che l'impegno e lo sforzo che tutti insieme abbiamo messo siano il segno più alto e più ampio di una presenza e di un vero *bipartisan* nella lotta alla criminalità organizzata, senza il quale ogni tipo di intervento dello Stato rischia di essere debole, minimale, inefficace. pertanto il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare e voglio ringraziare sinceramente tutti i colleghi Capigruppo per aver accolto la richiesta che noi abbiamo formulato di una corsia preferenziale per il provvedimento in esame che oggi, grazie a tutti noi, vedrà la luce.

tra importanti pezzi della società civile, le forze politiche, i Gruppi parlamentari. Quindi, per ragioni di merito, per quanto è stato già detto - e che condivido dagli altri esponenti dei Gruppi che sono intervenuti prima di me, ma anche per una ragione simbolica molto forte, che è stata sottolineata ed evidenziata anche dal senatore D'Alia, ossia il fatto che proprio oggi è importante che il Senato il Senato in maniera convergente approvi questo provvedimento che diventa anche un segnale, un elemento simbolico molto forte per dire che chi si muove sul terreno della legalità, chi è all'avamposto della legalità, soprattutto in alcune aree del Paese, merita la solidarietà operativa delle istituzioni, ed in questo caso del Senato della Repubblica attraverso l'approvazione di questo segnale

Presidente, anche noi abbiamo lavorato per il disegno di legge in esame, sia alla Camera che al Senato, con particolare convincimento. Non ritorno sui punti e sui limiti che alcuni colleghi hanno sollevato. Questo provvedimento interviene in un campo molto delicato, che attiene alla legalità e anche alla democrazia.

interviene su un tema molto importante: la legalità e la democrazia del nostro Paese e l'intreccio e il condizionamento politico-mafioso che sul voto si può esercitare e si è esercitato, come ci dicono tanti fatti, tante inchieste e tante indagini. Ci dicono, altresì, come tale condizionamento nei fatti rischia di diventare endemico in tanti territori del nostro Paese, e sicuramente non soltanto in quelli che fino adesso abbiamo considerato a forte infiltrazione mafiosa. Questo rapporto è da spezzare. È questa la vera battaglia democratica per restituire dignità alla politica e anche per liberare alcuni territori da una morsa che li stritola e che tende a perpetrare sottosviluppo, dipendenza e

Noi sappiamo che i soggetti di cui tratta il provvedimento, che sono dediti ad attività delittuose e spesso appunto di tipo mafioso, sono anche tali da controllare, attraverso la scelta di un candidato o di più candidati, il funzionamento, la vita e le scelte delle pubbliche amministrazioni. Questa ‑ a nostro avviso ‑ è la porta delle infiltrazioni criminali dentro le istituzioni. Questa è la connessione che lega concessioni di appalti, lavori pubblici e quanto altro conosciamo. Questo è anche il male oscuro e profondo del corrompimento delle nostre istituzioni. È un grimaldello che può minare profondamente la vita delle comunità e ‑ come si è dimostrato ‑ i legami e le catene delle filiere sono molto lunghi e molto più complessi del passato.

Il lavoro nella Commissione è stato lungo, e sappiamo che la larghissima intesa che si è ottenuta nasce proprio dalla consapevolezza che il traffico di voti, il condizionamento del voto di preferenza, che non a caso

Le mafie ormai non scelgono un partito, senatore Longo, ma credo lavorino sui candidati - come è dimostrato almeno fino a questo momento -, talvolta anche su più fronti e in tanti centri, come ci dicono anche alcune relazioni delle procure distrettuali che seguono soprattutto il flusso del denaro, per accrescere il loro potere sociale ed economico. È evidente, tuttavia, cari colleghi, che nessuna legge e nessuna pena potrà bastare, se non ritorna in campo la politica, o meglio una buona politica. Sicuramente dobbiamo interrogarci sulle modalità di costruzione del consenso in tante realtà, sul senso di responsabilità verso i cittadini quando esercitiamo la funzione di amministrativa sulla qualità della proposta politica e della rappresentanza degli interessi sociali. I principi invocati dall'articolo 97 della nostra Carta costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione non sono antiche parole nostalgiche,

Forse è solo su questa strada, con questo piccolo contributo di oggi, che possiamo sfuggire al qualunquismo e al populismo, che sono due facce della stessa medaglia. Forse possiamo tentare di restituire dignità alla politica,

Signora Presidente, riconfermando tutte le considerazioni rese in sede di discussione generale, condividendo quanto detto da tutti i colleghi intervenuti, rassicurati in modo particolare dalle parole del sottosegretario Davico, che impegna tutto il suo ufficio e il Ministero a sorvegliare attentamente questa materia così complessa,

con l'aggiunta del compiacimento che in tempi rapidi si giunga alla piena approvazione. Mi permetto di aggiungere anche il compiacimento per il voto unanime che converge su questo testo e il compiacimento perché la motivazione del voto favorevole che ho l'onore di rendere a nome del partito di maggioranza relativa è sostanzialmente consonante nei passi essenziali anche con quello che il maggior partito di opposizione poco fa ha reso a quest'Assemblea. Mi sembra un bel segno.

che abbiamo ingaggiato (consentitemi di utilizzare il verbo al plurale). Vero è che nessuna norma riuscirà ad esaurire questa battaglia o questa guerra ed è vero che la criminalità inventa sempre nuovi strumenti per aggirare, per inquinare, per eludere le norme. E assolutamente in argomento, poco fa proprio un autorevole collega ci ricordava che gli stessi dibattiti, ad esempio, in tema di moralizzazione del sistema elettorale e di buone tecniche nella individuazione del ceto politico elettivo si prestano a doppio taglio con le quali noi vorremmo, con la massima buona fede, vibrare i nostri colpi. Ed è sicuramente animato da buona fede chi parla di reintroduzione di un meccanismo di espressione delle preferenze nelle elezioni per favorire la trasparenza delle scelte e per reprimere o prevenire fenomeni di cortigianeria o dittatura dittatura dei partiti. Però è altrettanto vero, ed è assodato, che l'uso della preferenza è stato lo strumento essenziale di tutti i malcostumi e delle penetrazioni mafiose e malavitose di ogni genere un po' in tutta l'Italia e in particolare in alcune Regioni. Ma è pur vero che anche i sistemi, che pure da molti vengono auspicati, fondati su collegi uninominali riferiti a piccole porzioni del territorio e piccole comunità si prestano altrettanto a questo tipo di condizionamento e di inquinamento, se è vero che con 50, 100 o 200 voti manovrati da questo o quel soggetto poco raccomandabile si determina la vittoria o la sconfitta di un determinato candidato in una piccola parcella del territorio nazionale. Quindi si può dire, con tutto realismo, che stiamo varando una norma sicuramente doverosa,

Vere sono tutte le osservazioni fatte sia dal collega Li Gotti che dal collega Longo, e cioè che la normativa non riesce ad esaurire la complessa casistica ed è vero ancora - dobbiamo dircelo da giuristi, da persone che hanno il senso del diritto, dello Stato e delle garanzie - che i problemi sicuramente insorgeranno in sede di attuazione specifica si tratterà di applicarla ai casi concreti. Sarà ben difficile distinguere le manifestazioni di propaganda classicamente intese da quello che è un corri-voce, un passaparola, un presentarsi in ambienti ristretti e parlare facendo circolare la voce a sostegno o contro questo o quel candidato o gruppo di candidati.

ed avvertano la necessità di dimostrare, attuare, garantire e mostrare all'opinione pubblica la forza etica con cui sanno impegnare se stesse, non solo nell'individuazione delle candidature, ma anche nella messa in moto di tutti i meccanismi delle macchine elettorali, sapendo sottoporsi ad un giudizio trasparente ed inclemente, perché no, ma certamente rigoroso dell'opinione pubblica circa gli strumenti e le individualità capaci di mettere in campo nel momento supremo della verifica democratica che si sostanzia nelle consultazioni elettorali. Con questo auspicio, con questi sentimenti e con questa presa d'atto, a nome del Gruppo come episodio della determinata ed intransigente lotta contro la criminalità organizzata - versante su cui militiamo senza riserve e senza sottintesi - annuncio senz'altro il voto favorevole

Il baluardo contro l'invasione dell'Europa da parte dell'Islam ha avuto la meglio. Noi vogliamo ricordare questo giorno per dedicarlo alle tantissime vittime cristiane per opera di fanatici dell'Islam. Arshed Masih, come ricorderà certamente la Presidente, era un autista pakistano di fede cristiana bruciato vivo per essersi rifiutato di convertirsi all'Islam. La moglie, andata in caserma per denunciare la violenza, venne stuprata e torturata dai poliziotti davanti ai suoi figli. Questa non è affatto una storia di altri tempi:

Paese che tanto tiene ad entrare in Europa e dove in effetti prediligono ammazzare i nostri sacerdoti cristiani! Voglio soltanto ricordare ai colleghi che nell'ultimo secolo sono stati martirizzati ben 50 milioni di cristiani nel mondo: praticamente è scomparso un Paese grande quanto l'Italia.

delle persone musulmane praticanti che si sono convertite al cristianesimo. Inoltre, cosa ancora più grave, il Sudan è lo Stato che ha rimpiazzato gli Stati Uniti nella Commissione per i diritti umani nelle Nazioni Unite. Signora Presidente,noi

A Genova purtroppo si registra un disperso, un operaio di 44 anni di cui si sono perse le tracce, ma la situazione, che avete potuto verificare dalle immagini televisive, per chi l'ha vissuta sul territorio è veramente drammatica.

una distruzione del territorio veramente forte. Ricordo questi eventi nell'Aula del Senato perché, come certamente il Governo saprà, è già arrivato da parte del Presidente della Regione Liguria la richiesta dello stato di emergenza, e ovviamente di finanziamenti,

la possibilità di derogare al Patto di stabilità; oltre a questo, ovviamente, la possibilità di sospendere i tributi per quegli esercizi commerciali e quelle imprese che sono stati danneggiati dall'alluvione. Davvero l'urgenza è in questo caso assolutamente essenziale.

in cui i serbi bloccarono l'Islam a Kosovopoli; di lì in poi nacque un modo particolarmente cruento di difendere l'Europa giudaico-cristiana dalla presenza di musulmani, con la persecuzione nei confronti dei kosovari. se dobbiamo celebrare qualcosa, credo si debba celebrare l'impegno dell'Italia relativamente alle discriminazioni e alle persecuzioni nei confronti dei cristiani e quindi dare forza e magari qualche finanziamento in più ai nostri sforzi internazionali, piuttosto che una battaglia

per motivi non istituzionali, ma meramente politici. Il comma 2 dell'articolo 1 del Regolamento del Senato stabilisce che i senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

comportamenti o possedimenti di membri del Parlamento, ma anche per gravissimi fatti come l'attentato nei confronti del direttore di "Libero". All'inizio di questa legislatura ci siamo trovati di fronte ad una situazione quasi simile, relativamente alla Commissione di vigilanza RAI. Non vorrei che ancora una volta, ostaggio di diatribe di oligarchie partitocratiche, ci si dovesse trovare a non far funzionare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il presidente D'Alema ha convocato altre due riunioni per martedì e mercoledì; credo,

Signora Presidente, tra la CONSOB e le società quotate, soprattutto le banche, vi è un sistema di "porte girevoli", giacché provengono dalle banche

per essere designato dal gruppo Caltagirone nel consiglio di amministrazione dell'ACEA, società che ricade sotto la vigilanza della stessa CONSOB. Non la voglio fare lunga, ma sottolineo i mercati non aspettano i comodi del Governo, non aspettano che si metta fine ai litigi e al braccio di ferro tra il Ministro dell'economia e delle finanze

molto vicino, anzi sodale dell'ex presidente Cardia e con un passato nel settore bancario, non sembra in grado di andare oltre i meri annunci.

si faccia parte attiva per far sì che i due provvedimenti possano essere portati con celerità all'approvazione del Senato della Repubblica.

perché oltre all'attività dei Capigruppo anche la Presidenza possa intervenire sull'ordine del giorno in riferimento ad alcuni disegni di legge dei quali le Commissioni di merito hanno già completato l'esame e

di questo anno, visto che tutti i Gruppi si sono ritrovati attorno ad una proposta comune e a un testo unificato.